in oggetto, dalle notizie fornite dalla Direzione provinciale del lavoro di Lucca e dalla prefettura di Lucca è emerso quanto segue. In data 23 e 24 aprile 2007, due funzionari in servizio presso la Direzione provinciale del hanno effettuato un accesso ispettivo presso la sede della ditta FAPIM spa in Altopascio, allo scopo di verificare il rispetto, nei confronti del personale occupato, dei diritti costituzionalmente garantiti e delle norme legali e contrattuali di tutela dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda. Gli ispettori hanno riscontrato un atteggiamento collaborativo e di disponibilità da parte della direzione aziendale. Nel corso delle indagini sono state acquisite dichiarazioni di alcuni lavoratori, sei per la precisione. I lavoratori interpellati hanno fatto parte della RSU fino all'agosto 2006, data in cui la stessa è decaduta per effetto delle dimissioni volontarie della maggioranza dei componenti, dimissioni delle quali durante l'accesso non si sono apprese le motivazioni. Attualmente, non risulta alcuna proposta dei lavoratori per la costituzione di una nuova RSU. Nel corso dei colloqui con i lavoratori intervistati, non è emerso che l'azienda abbia frapposto ostacoli alla costituzione della prima RSU. I lavoratori intervistati dichiarano che a loro non risulta che la dirigenza aziendale sia mai intervenuta impedendo ai lavoratori l'iscrizione al sindacato o influenzando le scelte dei lavoratori. Agli stessi non risulta che la dirigenza abbia espresso valutazioni personali nei confronti di alcuno dei candidati RSU. Attualmente, su un totale di 437 dipendenti (di cui 71 a domicilio), risultano iscritti 42 dipendenti alla CGIL e sei alla CISL. Il Presidente della FAPIM spa dichiara di non aver mai effettuato, personalmente o tramite terzi, ai fini dell'assunzione, indagini sulle opinioni politiche e/o sindacali dei lavoratori occupati. I lavoratori intervistati riferiscono di non essere a conoscenza di episodi collegabili a discriminazioni perpetrate dall'azienda nei confronti di lavoratori e legate all'adesione al sindacato o alla partecipazione ad uno sciopero, seppure risulta che nell'anno 2000 fu indetto uno sciopero aziendale al quale parteciparono anche lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e alcuni di questi promossero una controversia giudiziaria contro la società, addebitando il mancato rinnovo contrattuale a tale adesione. Il tribunale di Lucca, con sentenza del 24 dicembre 2001, rigettò il ricorso asserendo la mancanza del nesso causale e la non sindacabilità delle scelte organizzative dell'azienda. Tra l'altro una dipendente, che nel 2000 aveva un contratto di formazione lavoro, ha riferito di avere partecipato allo sciopero e di essere stata assunta a tempo indeterminato. Risulta che in azienda vi sia stato un rapporto di legittima contrapposizione con le RSU che comunque sono state sempre ricevute dal Presidente del consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne abbiano fatto richiesta. Di ogni riunione viene redatto verbale sul quale vengono indicati gli argomenti trattati e le proposte risolutive. Copia dei verbali è stata acquisita nel corso delle ispezioni. Risulta che, ogni fine d'anno, nell'azienda si svolge un'assemblea durante la quale la proprietà illustra l'andamento dell'impresa attraverso i risultati di esercizio dell'anno in corso, gli investimenti in essere e le previsioni per gli anni a venire. I partecipanti hanno la facoltà di prendere la parola ed esprimere liberamente la propria opinione. I lavoratori intervistati hanno riferito che nel corso di tali riunioni non sono mai state affrontate questioni sindacali né che a loro risulti sia stato effettuato alcun sollecito nei confronti dei capireparto a redigere e sottoscrivere comunicazioni contrarie alle organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda lo spostamento di alcuni reparti in un altro stabilimento distante circa un chilometro e mezzo, agli intervistati non risulta ci siano state lamentele da parte dei lavoratori, anzi dalle dichiarazioni rese dagli stessi risulta che a seguito di detto trasferimento siano migliorate le condizioni dei lavoratori dei reparti anche con riferimento agli spazi e ai rumori. Relativamente al rischio ambientale e ai comitati composti dagli abitanti è emerso che il ricorso presentato dal comitato paesano al TAR è stato definito a favore della FAPIM. Il TAR, avendo ritenuto fondate le argomentazioni della società, ha concesso l'autorizzazione all'inizio dell'attività produttiva all'interno dello stabilimento già dal novembre 2006. Non è a conoscenza degli intervistati che i lavoratori abbiano raccolto firme in altre aziende sottoscrivendo una petizione da inoltrare alla prefettura di Lucca. Risulta loro che tale raccolta di firme è stata promossa dai rappresentanti provinciali CGIL e CISL fuori dai locali aziendali e le mille firme raccolte dalle organizzazioni sindacali appartengono a lavoratori di altre aziende della piana di Lucca. A nessuno è preclusa la possibilità di accedere ai locali della mensa aziendale la quale, infatti, risulta frequentata dalla maggioranza dei lavoratori ai quali viene elargito un contributo caffè e la relativa pausa non è registrata dall'azienda, che ha predisposto diversi "punti *break*" nei vari reparti. Nell'azienda si svolgono attività di "turnisti" e "a giornata". I turnisti usufruiscono di trenta minuti per la pausa pranzo e dalle interviste risulta che rimane nella loro libera scelta se consumare il pasto a mensa o rimanere sul

Lo straordinario, che prevede una maggiorazione della normale paga oraria, viene equamente distribuito e puntualmente retribuito. La legge antinfortunistica viene rispettata, periodicamente vengono tenuti corsi di aggiornamento per il personale e l'azienda ha investito in impianti di alta tecnologia che riducono il rischio infortunistico. Gli infortuni occorsi sono stati indennizzati dalla società ed, effettivamente, come rappresentato nell'interrogazione, un infortunio è stato addebitato a colpa della società ed il Presidente del consiglio d'amministrazione è stato condannato a risponderne penalmente. E' altrettanto vero che la società ha in corso una causa per *mobbing* pendente innanzi al tribunale. I lavoratori intervistati hanno riferito un'apertura dell'azienda nei confronti delle RSU, ma una totale chiusura nei confronti delle organizzazioni sindacali territoriali. Però, il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali provinciali per condotta antisindacale si è concluso con sentenza n. 477 del 24 aprile 2001, con la quale il tribunale rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Ha trovato riscontro quanto evidenziato nell'interrogazione 3-00573 ed è evidente che il comportamento aziendale testimonia un conflitto aperto con il sindacato territoriale, specie per quanto attiene alla lettera di accompagnamento. Si ritiene che la circostanza della divulgazione al personale del contenuto dell'interrogazione parlamentare, tuttavia, essendo atto pubblico, non costituisca in sé condotta antisindacale. Con riferimento, poi, ai comportamenti antisindacali descritti e alla richiesta di iniziative da parte del Ministero, si evidenzia che allo stesso non è istituzionalmente conferito un potere di intervento diretto in proposito, né un potere di coercizione nei confronti del datore di lavoro. Il rispetto delle norme dello Statuto dei lavoratori e la conseguente repressione dei comportamenti datoriali di carattere antisindacale (configurabili come diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero), possono essere invece efficacemente attuati, come è noto, in sede giudiziale, attraverso lo speciale strumento di tutela previsto dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970. In particolare, il predetto articolo prevede un procedimento di rapido svolgimento, il cui provvedimento finale è immediatamente esecutivo. La norma stabilisce che legittimati ad agire sono gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, i quali possono proporre ricorso alla magistratura del lavoro del luogo ove vengano posti in essere i comportamenti antisindacali. Il giudice, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro con decreto motivato immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. In conclusione, conclusione, avendo l'accesso ispettivo riguardato l'intervista ad un esiguo numero di dipendenti e laddove venisse richiesto un ulteriore approfondimento, si dichiara fin d'ora la disponibilità ad adoperarsi in tal senso.

cui l'azienda è - come hanno detto? - collaborativa e responsabile e in cui in questi anni non è accaduto niente.

se è proprio vero che questo è un paradiso terrestre. La ringrazio molto della clausola di salvaguardia finale, quando ha detto: se su 437 dipendenti se ne sono sentiti sei, forse

nel mese di agosto dell'anno scorso sei rappresentanti (la maggioranza) delle RSU si sono dimessi contemporaneamente.

Può non presentarsi? Immagino di sì. Denota questo uno spirito di collaborazione istituzionale e sindacale? No. Se io fossi in

Non è per caso che essi sono stati fatti alla presenza - per carità, collaborativa e responsabile, si intende - dell'azienda? Non è che che questi lavoratori sono stati costretti - e sottolineo costretti - a parlare in presenza di questa illuminata direzione aziendale? È vero

Vi sono molte lavoratrici operate di tunnel carpale che magari possono anche non protestare per un elemento di intimidazione, ma gli interventi chirurgici che hanno dovuto subire sono reali. Queste patologie sono dovute ai ritmi di lavoro. L'Ispettorato del lavoro si interroga su tali questioni o fa finta che non succeda niente? E chi è che dovrebbe discutere come sono organizzati i ritmi di lavoro, verificarne l'idoneità, se non il sindacato, che è costantemente escluso, come del resto lei ha detto e come le è stato riferito? Il Presidente del consiglio d'amministrazione di una azienda grande, non solo per una zona come quella di Lucca ma in generale, che ha quasi 500 tra addetti diretti ed indiretti, è stato condannato a cinque mesi di reclusione per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e viene detto nell'informativa che vengono rispettate tutte le norme di sicurezza. Ci sono stati degli infortuni, l'ultimo dei quali con sette mesi di prognosi. L'Ufficio del lavoro di Lucca si interroga su queste modalità? Al Ministero del lavoro vi interrogate sul fatto che la FAPIM è l'unica azienda, per lo meno della zona, dove non esiste alcun contratto di secondo livello, così come previsto dalle norme che regolano la materia? E non è forse vero che è compito della contrattazione aziendale lo stabilire il rispetto delle condizioni normative di sicurezza, gli investimenti e via discorrendo?

il paradiso terrestre, dove i rapporti di lavoro tra direzione e operai sono talmente idilliaci che essi a fine anno si riuniscono, l'azienda presenta bonariamente i risultati conseguiti, gli investimenti e ognuno ha la possibilità di parlare (e immagino,

si dovrà mettere in discussione il modo come si lavora e le informazioni che vengono fornite a lei, e tramite lei, al Parlamento, perché poi di questo si tratta. Su tali informazioni, ovviamente, noi svolgeremo nuovamente

notizie fornite - della risposta che lei ci ha dato, che ci lascia completamente insoddisfatti e, come dicevo all'inizio, un po' sgomenti per il modo in cui tali risposte vengono preparate.

sulla base delle notizie fornite anche da Terna S.p.A., si osserva che nel periodo estivo 2006, il sistema elettrico italiano, in base alle valutazioni previsive sullo stato dello stesso, effettuate nei mesi precedenti, presentava una situazione complessiva non preoccupante. La riprova che la situazione non fosse critica si è avuta il 27 giugno 2006 quando si è registrata la punta estiva con un fabbisogno complessivo pari a 55.619 Nonostante l'incremento dei consumi rispetto all'anno precedente nel giorno di massima punta, vi era un margine di riserva adeguato a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico italiano, senza quindi la necessità di approntare alcun tipo di intervento. A partire da lunedì 24 luglio 2006 e nei giorni successivi, si è verificata tuttavia una situazione di carenza di energia elettrica che ha interessato tutta l'Europa. La situazione di criticità è stata determinata da condizioni climatiche eccezionali che hanno incrementato i consumi e ridotto le capacità produttive delle centrali di vari Paesi, come dimostrato dalle tensioni di prezzo registrate in quei giorni su tutte le Borse europee dell'energia. In Italia, nei giorni 25, 26 e 27 luglio 2006, si è registrata un'elevata domanda di energia, una forte riduzione delle importazioni e, contestualmente, un consistente incremento dell'*export* di energia, a cui si sono aggiunti eventi eccezionali quali avarie di alcuni impianti in misura superiore alla media ed un incremento, rispetto ai valori *standard* stagionali, del numero di impianti di produzione disponibili che hanno garantito una capacità produttiva inferiore rispetto alla loro capacità nominale. In ragione delle criticità evidenziate, il sistema energetico nazionale non disponeva di adeguati margini di riserva di energia nelle ore di maggiore utilizzo. Al fine di garantire la copertura del fabbisogno, sono state adottate tutte le misure necessarie, quali il ricorso alla riserva esistente e ad acquisti di energia nelle borse europee. In particolare, Terna S.p.A., in qualità di concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento, in virtù del decreto ministeriale 20 aprile 2005, ha provveduto a massimizzare l'utilizzo della capacità produttiva disponibile in Italia e ad acquistare l'energia disponibile sui mercati europei per reintegrare, almeno parzialmente, la riduzione delle importazioni. Nonostante gli acquisti dall'estero di quantitativi di energia, nell'esercizio in tempo reale non vi erano adeguati margini di riserva nelle ore di maggiore utilizzo e Terna, quindi, ha dovuto provvedere all'interruzione della fornitura di energia elettrica ai soggetti titolari di contratti di interrompibilità, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dalla normativa vigente e dai contratti stipulati da questi soggetti, al fine di evitare maggiori rischi per il sistema. Il distacco della fornitura è avvenuto, pertanto, solo nei confronti dei clienti interrompibili, ovvero di quei soggetti industriali che volontariamente hanno fatto richiesta di prestare il servizio di interrompibilità, alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo economico per tale servizio, e non nei confronti dell'utenza diffusa. Ciò premesso, vale la pena sottolineare come il sistema elettrico debba essere in condizione di equilibrio istantaneo tra domanda ed offerta, non potendo, come è noto, immagazzinare energia. Per questi motivi, è possibile che vi siano disponibilità di energia da esportare in determinate ore del giorno e, nello stesso periodo, carenza di offerta nelle ore di punta tale da motivare il ricorso al servizio di interrompibilità. Per quanto riguarda i temi legati alla tutela dei consumatori, si ricorda che con il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (il cosiddetto decreto Bersani), di recepimento della direttiva comunitaria 96/92/CE, è stata avviata la riforma strutturale del settore elettrico in Italia. Tale decreto ha segnato l'inizio del processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica svolte nel rispetto degli obblighi derivanti dal servizio pubblico. Successivamente, con la direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (che abroga la precedente direttiva 96/92/CE), sono state introdotte una serie di misure per l'apertura completa del mercato dell'elettricità a vantaggio del consumatore europeo. La direttiva mira al rafforzamento delle condizioni favorevoli ad una concorrenza leale ed equa ed alla realizzazione di un autentico mercato unico. Essa impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per realizzare puntuali obiettivi tra cui anche la protezione dei consumatori vulnerabili, la tutela dei diritti fondamentali e la coesione economica e sociale dei consumatori. Il Governo, con il disegno di legge Atto Senato n. 691, contenente disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno 2006 ed attualmente in corso di esame al Senato presso la competente Commissione parlamentare, intende recepire nell'ordinamento italiano la suddetta direttiva In particolare, viene stabilito il principio di indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica concernenti la sicurezza e l'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture nonché l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive che fornirà il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, viene previsto che sia garantita l'offerta di energia elettrica a condizioni di mercato ai clienti degli ambiti territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato. Ancora, è prevista la promozione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica tenendo conto dell'esigenza di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento oltre che, naturalmente, della sostenibilità ambientale. Tali misure, favorendo il meccanismo della libera concorrenza su cui poggia la liberalizzazione, porteranno dei vantaggi per i consumatori, promuovendo forniture più economiche, flessibili e di qualità, traducendosi in maggiore efficienza sul costo di produzione di energia elettrica con dirette conseguenze sulla componente tariffaria direttamente legata a quest'ultimo. In merito alla garanzia di fornitura, si osserva che ad Aquirente Unico S.p.A. è affidato il compito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 di assicurare la fornitura di energia elettrica, a prezzi competitivi e in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, ai "clienti vincolati", in modo da consentire anche a tali consumatori di beneficiare dei vantaggi del processo di liberalizzazione del settore. Anche dopo la completa apertura del mercato ai clienti oggi "vincolati", fissata al 1° luglio prossimo, i consumatori continueranno a beneficiare di un sistema di garanzia (fornitore di ultima istanza) in grado di assicurare l'universalità e la continuità del servizio. Si sottolinea, quindi, la necessità che il disegno di legge delega, oggi all'esame del Parlamento, venga approvato in tempo utile per l'esercizio della delega prevista e per la concreta definizione di tali forme di garanzia. Vorrei aggiungere che, in riferimento a temute situazioni di criticità per i mesi estivi, è già operativo da circa due mesi un comitato che vede la partecipazione non solo del Ministero dello sviluppo economico e del Dicastero dell'ambiente e delle Regioni interessate, delle autorità di bacino interessate e dei consumatori industriali, elettrici ed agricoli per attivare, come in effetti è già accaduto, delle procedure virtuose, tanto da limitare in questa fase l'uso idroelettrico e preservare risorse preziose per eventuali situazioni di criticità che dovrebbero e potrebbero, sulla base di valutazioni previsive, verificarsi nel corso dei mesi più caldi. in atto, anche in una congiuntura e con strumenti di natura congiunturale, l'attenzione necessaria per ridurre al minimo i disagi per gli utilizzatori, in questo caso, in modo particolare per il sistema produttivo, dal momento che la priorità per gli utenti civili viene puntualmente confermata. Signor Presidente, signor Sottosegretario, la ringrazio per essere venuto qui oggi a rispondere a questa interrogazione, che è datata

quasi drammaticamente attuali: il primo è quello relativo all'informazione del consumatore e l'altro, invece, è di merito e concerne la potenzialità del nostro sistema di produzione e distribuzione dell'elettricità. problema dell'informazione è quanto mai sconcertante, perché evidentemente vengono passate ai mezzi d'informazione notizie che sono assolutamente diverse dalla realtà. Infatti, se è vero come è vero, che in alcune situazioni può esserci anche un'esportazione di energia, è altrettanto vero che noi siamo un Paese importatore di energia e di materie prime per la produzione di energia. Quindi, diventa difficile dipingere, come è stato fatto e come ho ricordato nell'interrogazione, un'Italia

Allora, questa è un'informazione distorta, che crea grande confusione nei nostri concittadini. Infatti, il nucleare è una fonte di energia straordinaria pulita se viene prodotta fuori dai confini nazionali; è una fonte straordinaria e necessaria se viene importata. Peccato che tutto questo comporti due grossi problemi

considera che la Francia, che è uno dei nostri grandi fornitori, paga l'energia elettrica circa 30 euro a megawatt, si accorgerà quanto il consumatore debba pagare per questa fornitura.

per quattro elettrodotti; più di tanta energia non riusciamo a trasportare. Allora, capisco che il Governo, in questi giorni di allarme, abbia detto ai consumatori

Mi pare una risposta che meriterebbe di essere commentata ovvero meriterebbe ben altri interventi, come quello, che auspico, di un nuovo Piano energetico nazionale.

in modo particolare, si pone un problema di compatibilità. Rispetto a ciò, è noto che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il consiglio d'amministrazione dell'ENEA è composto dal Presidente e da sette membri, in possesso questi ultimi di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due designati dal Ministero dello sviluppo economico, due dal Ministero dell'università e della ricerca, due dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2006. Con la trasparenza che contraddistingue l'azione del Ministero e della quale l'interrogante dà atto riferendo sulla collaborazione concretamente offerta per le informazioni richieste, si risponde ai punti sollevati nell'interrogazione stessa. L'interrogante si sofferma tra l'altro su una presunta commistione di ruoli tra vigilante e vigilato a proposito della nomina nel consiglio di amministrazione di due dirigenti generali del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, si fa osservare che le ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere d'amministrazione dell'ENEA sono espressamente previste e disciplinate dall'articolo 111 del decreto ministeriale n. 165 del 2006, recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. Nessuna di esse ricorre nel caso di specie; in particolare, il ruolo di dirigente generale del Ministero esula sicuramente dalla «carica di Governo» di cui al 1° comma della citata disposizione, attesa la cesura realizzata dal decreto legislativo n. e successive modifiche e integrazioni, tra attività d'indirizzo politico-amministrativo, spettante all'autorità politica, e quella gestionale in senso stretto, di competenza esclusiva dei dirigenti. Tale netta separazione è stata da ultimo ribadita dalla legge n. 215 del 2004, che ha circoscritto l'operatività del conflitto di interessi alla titolarità di cariche politiche di Governo. Tanto a prescindere dal fatto che nel caso non sono ravvisabili le condizioni per l'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto di interesse. La stessa natura di ente strumentale dell'ENEA, istituzionalmente chiamato a perseguire compiti propri e esclusivi del Dicastero, esclude per definizione la sussistenza in capo al dirigente generale per l'energia, dell'eventuale «conflitto di interessi non occasionale», cui fa cenno l'ultimo comma del citato articolo 111. Né risulta violato, nel caso di specie, il principio di «buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione» *sub* *specie* di dualità soggettiva controllore-controllato. Invero, l'articolo 22 del decreto legislativo n. 257 del 2003, recante riordino della disciplina dell'ENEA, affida la vigilanza sull'andamento dell'ente in parola e sul perseguimento dei relativi fini istituzionali al Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), in relazione a prerogative di organo d'indirizzo politico-amministrativo, indicando, nel contempo, gli atti soggetti all'approvazione. Trattasi, peraltro, di atti la cui adozione deve ricondursi all'iniziativa del direttore generale dell'ente e alla successiva approvazione del consiglio. In buona sostanza, il consiglio d'amministrazione dell'ENEA, come fatto palese dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 2003, non ha poteri gestionali in senso stretto, ma di programmazione, indirizzo e controllo strategico. La presenza di alti dirigenti del Ministero in seno a tale collegio non realizza alcuna indebita commistione tra controllori e controllati. Diversa conclusione s'imporrebbe se un soggetto stabilmente incardinato nella struttura ministeriale fosse chiamato a rivestire l'incarico di Direttore generale, in quanto dotato di effettivi poteri gestionali, come disciplinato dall'articolo 12. Ne è riprova la circostanza per cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 gennaio 1996 di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, espressamente sancisca l'incompatibilità della carica di Direttore con qualsiasi impiego pubblico e privato. La stessa presenza consente, per contro, di realizzare quel collegamento strutturale tra soggetto designante e organo collegiale dell'ente controllato, che garantisce la rappresentanza del primo nel secondo così come testualmente sancito dalla Corte dei Conti con l'atto 1869 del 18 giugno 1986. Non può peraltro sfuggire che il Ministro dello sviluppo economico, nell'esercitare il potere di designazione al medesimo espressamente conferito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 2006, si è scrupolosamente attenuto al principio per cui «ove il potere sia dalla norma genericamente conferito, la scelta dei componenti degli organi collegiali degli enti controllati in rappresentanza di un dicastero deve cadere su soggetti stabilmente e organicamente in esso inquadrati ed in particolare sui dirigenti, cui tale funzione di rappresentanza spetta quale compito normale», anche questa è una citazione di un atto della Corte dei conti. Da parte dell'interrogante si sostiene, ancora, che la dottoressa Maria Cristina Battaglia e l'ingegnere Simone Molteni, rispettivamente nominati consiglieri d'amministrazione dell'ENEA su designazione del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente, non avrebbero «esperienze» gestionali, come richiesto dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 2003. L'articolo 6 parla di «competenze» gestionali e non di «esperienze», con ciò puntando alle «competenze» proprie di ogni percorso di studio applicato ad una esperienza professionale qualificata anche sul piano gestionale; una formulazione letterale quindi di ampio respiro, aperta a quegli stimoli innovativi che anche sul piano gestionale possono emergere nelle dinamiche della società e del mercato, senza per questo voler negare rilievo ai trascorsi lavorativi. Inoltre, la competenza gestionale deve essere considerata in relazione a materie differenziate, per le varie gamme di attività tecniche dell'ENEA. Dai *curricula* risulta che la scelta dei competenti Ministeri è ricaduta su persone che, in possesso di un bagaglio conoscitivo in materie rilevanti, hanno dimostrato anche competenze gestionali. Nel caso della dottoressa Maria Cristina Battaglia ciò emerge dai riferimenti all'esercizio di responsabilità di coordinamento di area tecnico-scientifica dell'INFM, alla Presidenza di Sviluppo Italia Liguria, a pubblicazioni con approfondimenti su problemi gestionali e su applicazioni ad attività d'impresa, oltre che da una considerazione del complessivo profilo formativo. Nel caso dell'ingegnere Simone Molteni, ciò emerge dai riferimenti a responsabilità di direzione di progetti ambientali e ai mirati profili formativi sul tema dell'integrazione di *management* e tecnologia, con doti anche in gestione di relazioni in diverse lingue. Altre considerazioni dell'interrogante riguardano i mancati inserimenti nel Consiglio di persone con «esperienza» in campo nucleare ed in attività di ricerca. A parte che è lo stesso interrogante a dare atto di esperienze in tema di ricerca da parte dei consiglieri citati e senza inoltrarsi nelle specificità di altri organismi chiamati ad operare nel campo nucleare, è da dire che non si può comunque considerare il consiglio d'amministrazione come la sede di un confronto tra portatori di esperienze lavorative; occorre invece proiettare le professionalità, e non le mere «esperienze», dei soggetti in funzione delle esigenze proprie del ruolo istituzionale di tale organismo che è propriamente quello di disegnare gli indirizzi e le strategie dell'Ente. Partendo da questa diversa prospettiva, è chiaro come sia pienamente funzionale - e quindi corrisponda ad esigenze di ottimale amministrazione da parte del Ministero designante - individuare per il ruolo di componenti del consiglio d'amministrazione proprio i soggetti in grado di dare un «valore aggiunto» al perseguimento dei fini dell'ENEA, quale ente strumentale, tenendo conto, per le ragioni già esposte, delle professionalità rivestite in ambito ministeriale, come nel caso dei due direttori generali designati da questo Ministero, o dei percorsi individuali di professionalità e formazione.

dottoressa Rosaria Romano, prendo atto di tutte le complesse argomentazioni che il sottosegretario Bubbico ha prospettato riguardo la non presenza di un conflitto d'interesse tra questa posizione e la posizione di controllore in quanto direttore generale del Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, segnalo che il consiglio d'amministrazione, tra l'altro, elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente, approva il piano triennale, il piano annuale di attività, attività, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento. Tutte queste azioni sono poi ulteriormente soggette ad approvazione da parte del Ministero. Pertanto, sono le stesse persone che, da un lato, nel consiglio d'amministrazione partecipano all'approvazione di questi documenti e, dall'altro, in sede di Ministero vigilante, riscontrano la correttezza degli stessi. Non mi sembra che sia il massimo. Devo riscontrare che, nella mia esperienza di cinque anni al MIUR, il ministro Moratti ed io stesso abbiamo sempre evitato questo tipo di posizione. Circa poi la responsabilità della designazione di due persone molto giovani

all'articolo 6 prevede esplicitamente che siano in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali»; non di competenze scientifiche e gestionali, ma elevate competenze. Lei, sottosegretario Bubbico, non ha mai menzionato questo aggettivo che è qualificante: le competenze gestionali devono essere elevate. Ora, non si può francamente dire che chi si è laureato nel 1998 o nel 1999 ha avuto modo di fare un'esperienza gestionale di tipo elevato; né gli studi (uno laurea in fisica, l'altro laurea in ingegneria edile) hanno avuto modo di sviluppare questa competenza, perché sono due lauree tecniche. Pertanto, non ci sono elementi, salvo quelli naturali: i giovani sono brillanti e si faranno certamente e auguro loro una strada ricca di soddisfazioni; non mi si venga a dire però che posseggono già *ex ante* elevate competenze gestionali. In ultimo, mi consenta, signor Sottosegretario, di rinnovare la critica alla carenza di competenza specifica in ordine alle materie che il consiglio d'amministrazione dell'ENEA deve deliberare. Ripeto, questo consiglio d'amministrazione deve deliberare su materie di straordinaria complessità tecnico-scientifica, quali la fusione nucleare, i nuovi sviluppi dei reattori nucleari. In particolare, ricordo che (articolo 6) il consiglio d'amministrazione è competente per individuare gli obiettivi e le priorità delle attività dell'ente, per verificare l'attuazione dei programmi, e così via. In sostanza, ritengo che complessivamente le competenze delle persone che sono attualmente presenti nel consiglio d'amministrazione dell'Ente, per la loro esperienza, per la loro qualifica,